nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

sinceramente sono ancora alquanto perplesso per la non risposta del Vice Ministro sul problema delle delle birrerie artigianali, su un articolo imposto alla Camera e non si capisce da chi, non voluto da alcuna delle organizzazioni o dalle aziende che producono birra (anzi, con la loro contrarietà, stante la difficoltà di definire il concetto di birreria artigianale). di un articolo sospetto che sembra nascondere qualcosa di poco serio, come purtroppo avviene spesso nel nostro Paese. Non c'è stato verso si è deciso di non abrogare questo articolo misterioso. Certamente resto meravigliato ed esterrefatto, perché ciò poi si collega a tutto quello che viviamo in generale.

di sicurezza fatta dal Poligrafico dello Stato prevede che tanto hai acquistato e tanto puoi trasformare. Non c'è mai risposta e si continua a tacere su questo argomento

sebbene un'operazione di questo tipo porterebbe occupazione all'interno di un'industria di Stato. Porterebbe ricchezza alle casse dello Stato e farebbe chiarezza, innanzitutto, alla vittima vera di tutto questo, il consumatore, che non sa assolutamente ciò che mangia. Anche la

anche il confronto con gli altri. Si tratta di un problema serio. Rispetto a tutto quello che diciamo e facciamo, ma di che cosa stiamo parlando? Ci prendiamo in giro da soli? Facciamo dei piccoli passi in avanti, ma rispetto al grande tema non ci siamo. soluzioni. Non tuteliamo i consumatori, non tuteliamo lo Stato italiano, non tuteliamo le industrie di Stato italiane. E basterebbe così poco. Non è la fine del mondo. Vuol dire cozzare contro mondi

si ingrassano sempre di più e i loro prodotti non vengono mai toccati, neanche dall'aliquota IVA. Questa è la realtà. E al Governo si chiede di essere più forti e duri nel difendere ciò che è nostro, e non per una pretesa, ma perché è giusto che sia così.

perché ci rendiamo conto di tante questioni. Abbiamo sempre votato a favore, anche negli anni scorsi. Hanno votato a favore i nostri colleghi della Camera, ma evidentemente sono molto male informati

Quindi concludo confermando il voto di astensione.

l'azione del Governo sugli emendamenti. Gli emendamenti sono stati sostanzialmente tutti respinti, e non perché non validi nel merito - come dichiarato dallo stesso Vice Ministro, palesemente in imbarazzo nel dare qualche parere contrario

il Ministro ad avere maggiore pudore prima di andare in televisione a dichiarare che questo è l'esempio del malfunzionamento del bicameralismo perfetto. Questo, invece, è il perfetto esempio di come il Governo Renzi, a seconda della convenienza, acceleri su alcuni provvedimenti e li chiuda in qualche settimana.

tirandoli in lungo, in modo tale che a ogni elezione si possa andare dagli agricoltori facendo vedere che si sta facendo un passo in avanti, procrastinando la possibile soluzione ai problemi, ribadisco ancora una volta, caro Ministro di carta: attenzione, si può ingannare tutti una volta, qualcuno qualche volta, ma non si possono ingannare tutte le persone per sempre. E gli agricoltori, caro Ministro di carta, ormai hanno capito che l'agricoltura non è argomento importante e prioritario nelle politiche del Governo. Da cosa lo hanno capito? Lo hanno capito - ad esempio - dal fatto che in Commissione europea, o meglio a Bruxelles, non ci va lei, Ministro assente, a contrattare con gli altri *partner* europei o con il Governo di Bruxelles in merito alla difesa del *made in Italy.* Ci va il ministro Calenda a parlare di CETA - ricordo che è l'accordo tra l'Unione europea

Quindi ci siamo rassegnati a questo modesto collegato all'agricoltura. Anticipo già che il nostro voto non sarà favorevole, ma non sarà neppure contrario. Non può essere contrario perché ci sono passaggi importanti e utili, seppure in un ritardo di cui avete responsabilità. Ma non può certo essere favorevole, perché non vogliamo avallare il vostro modo di fare che utilizza l'agricoltura per il solo scopo elettorale, dimenticandone realmente i problemi. Non si fa fatica ad andare sul *web*, signora Presidente, a trovare, oltre al sito del Ministro dell'agricoltura, ben patinato e preciso, con interviste inginocchiate di domande e risposte in cui tutto va bene e funziona, anche dei commenti di agricoltori,

che si alzano al mattino e vanno a letto la sera e, dopo una giornata di lavoro, sanno che un vitello vale come un quintale di concime. Di questo stiamo parlando.

nascosta tra lo sport e la cronaca rosa, o non c'è per niente. Questo non è corretto, perché vuol dire nascondere alla conoscenza dei cittadini trattative che sono intimamente connesse con la difesa del *made in Italy*.

restano esposti per milioni di euro, dovendo pagare addirittura sanzioni dell'1 per cento perché sono in ritardo nella presentazione di documentazione, e non per colpa loro ma di AGEA? di AGEA? Ribadisco: basta andare a guardare sui siti. Mi sono fatto forte e sono entrato nel sito istituzionale del ministro Martina. In una intervista inginocchiata che gli è stata fatta qualche mese fa, il 23 maggio 2016, il «ministro di carta» Martina, alla domanda: «Pavia, provincia risicola. A che punto è la vicenda della clausola di salvaguardia che dovrebbe frenare l'importazione di riso indica dal Sud-Est asiatico?», risponde: «Abbiamo

«Lo abbiamo ribadito ai tecnici della Commissione che nei giorni scorsi sono stati a Castello d'Agogna. Ora ci aspettiamo di più dalla Commissione UE, perché le risposte arrivate fino ad ora sono insoddisfacenti». Immagino che alla lettura di questo commento del Ministro a Bruxelles siano tremati di paura e tremino ancora adesso come foglie. Non ce la fanno più dal terrore che il ministro Martina

e mozioni approvate in Parlamento, che poi non trovano attuazione nella realtà. Su dette cose si difende l'agricoltura nazionale, l'agricoltura del Paese, che in questo caso corrisponde anche all'ecosistema del territorio.

all'inaugurazione del 262° anno accademico dell'Accademia dei Georgofili, la relazione che si intitola: «Un grave errore demolire l'agricoltura».

riguardo all'embargo alla Russia. Si può parlare di collegato agricoltura, di interventi per mitigare i costi per l'agricoltura, le tasse, annessi e connessi. Per l'amor di Dio, piantatela con la storia dell'IMU, perché prima mettete le tasse, poi le togliete, e poi vi volete anche prendervi i meriti per averle tolte dopo aver creato danni agli agricoltori e agli altri cittadini

fate togliere le sanzioni alla Russia, perché la nostra agricoltura ne ha un grave danno. Su questo si misurano la qualità, l'azione e la forza del Governo, e non prendendo e mettendo un Ministro sulla carta stampata.

mio intervento in discussione generale con il seguente appello: vogliamo partecipare responsabilmente al futuro dell'agricoltura italiana. Abbiamo presentato diversi emendamenti, alcuni dei quali sono stati ritirati per non intralciare il lavoro che è stato fatto.

che autorizza le organizzazioni professionali di categoria alla

ma ancora una volta ribadisco che un ordine del giorno non si nega a nessuno, signor rappresentante del Governo. Soprattutto avevamo aspettative per quanto riguarda il riordino e la razionalizzazione degli enti

come quelli che ho citato, ma ce ne sono ancora altri. Penso - per esempio - alla soppressione durante la lettura alla Camera del reato di contraffazione alimentare. Lo avete tolto. Veramente non si capisce ancora perché. Avete annullato tutto l'articolato che riguarda la pesca e l'acquicoltura. Abbiamo tentato in tutti i modi di poter collaborare con il Governo, ma nulla. Bisognava andare avanti e basta. Avete

Bisogna capire quale nuovo modello di agricoltura vuole adottare il Governo per confrontarsi nel mondo e con tutti gli altri Paesi con cui siamo in competizione.

l'unico comparto che tira e produce fatti positivi per l'economia del nostro Paese. Ve ne siete vantati, ma non ne sono convinto come voi, perché l'agricoltura ha molto bisogno di interventi specifici e razionali e non raffazzonati, come tante volte è successo in questa legislatura. Vorrei parlare dei giovani.

I giovani imprenditori agricoli di oggi chi sono? Vorrei che facesse anche un'attenta verifica.

professionisti di buon livello che hanno sposato l'agricoltura. Questi sono i giovani che si affacciano al mondo imprenditoriale agricolo.

trascrizione agevolata dei trasferimenti per accorpamenti aziendali anche per imprenditori agricoli professionali,

magari iscritti all'albo degli avvocati o degli ingegneri, che hanno deciso di sostenersi attraverso il sistema agricolo,

che consentiva ai giovani imprenditori agricoli, per gli accorpamenti di azienda, di non pagare la cosiddetta tassa di trasferimento. Era stata concessa una tassa di trasferimento agevolata, che oggi è scomparsa. Ma volete ancora sciacquarvi la bocca a parlare di giovani imprenditori agricoli? Perché non date risposte in tal senso? Sto parlando di cose concrete e non del libro dei sogni. Lì bisogna dunque incidere, se si vuole aiutare l'imprenditoria agricola giovanile, anche professionalizzata dal punto di vista scolastico. Si tratta di una grande risorsa per il Paese, di una grande opportunità. Agevoliamo questi giovani!

mio intervento, signora Presidente e signor Vice Ministro. Questa è una grande opportunità perduta. Speriamo che ce ne sia qualche altra.

e non solo produce alimenti, ma è anche importante per la salvaguardia ambientale e per la valorizzazione turistica, soprattutto nelle nostre zone. Molti colleghi, nel corso della discussione generale, hanno sottolineato l'attenzione ai settori emergenti, a cominciare da quello del luppolo e delle birre artigianali,

in parte razze in pericolo di estinzione, ma sono una componente importante della biodiversità - affinché esse e le loro associazioni di allevatori abbiano anche in futuro l'attenzione, il rispetto e l'aiuto da parte del Ministero e non vengano affossate, perché non di rilevanza nazionale. Per i nostri territori questi piccoli allevatori svolgono un'attività di conservazione, di grande tutela per l'ambiente e di cura del suolo. Sono previsti, in ogni caso, passi positivi per la valorizzazione del marchio e per la competitività. Tuttavia, questo è un provvedimento che conferisce ancora una volta una delega molto forte al Governo su tutta una serie di punti cruciali. La delega è un'espressione di fiducia e di buona volontà da parte delle Camere circa la capacità del Governo di mettere in campo norme in grado di fare gli interessi del settore. I precedenti non sono sempre confortanti. Troppe volte, in vari settori, le leggi delega hanno creato nuova burocrazia per le aziende, che invece oggi avrebbero bisogno di una forte semplificazione normativa. questo vale soprattutto per le piccole e piccolissime aziende agricole, che sono il cuore pulsante dell'agricoltura di montagna. In questi anni, troppe volte ho visto che non si comprende soprattutto a livello ministeriale, la funzione dei piccoli agricoltori, che non è solamente economica, ma riguarda - lo voglio ribadire - anche la tenuta sociale di territori montani e svantaggiati, la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attrattività paesaggistica. Penso - ad esempio - alla norma contenuta nell'ultimo disegno di legge di stabilità, fortunatamente eliminata, che tentava di introdurre una serie di obblighi di gestione fiscale per le aziende con meno di 7.000 euro di fatturato annuo. Un'azienda che fattura meno di 7.000 euro all'anno è un'azienda che, nei fatti, non produce utili economici, ma fa un'azione di presidio del territorio, anche dal punto di vista ambientale e sociale, e tanti piccoli agricoltori creano diversità sia di prodotti sia di servizi. Il grande tema, allora, è come si aiutano queste aziende, come si stimola la nascita di consorzi di produttori; come, cioè, si mette a valore un sistema che dà vita alle produzioni qualitativamente più interessanti e che rappresenta anche un veicolo formidabile dal punto di vista del *brand* e del turismo. Dobbiamo salvaguardare la piccola proprietà contadina: la loro attività è il fondamento di una agricoltura praticata con entusiasmo. Ci sono ancora grandi margini per semplificare e ridurre quella burocrazia che, troppo spesso, è un ostacolo per la crescita e lo sviluppo del settore.

- prevede che ogni persona che detiene anche solo un alveare debba fornire comunicazione all'anagrafe apistica nazionale, con sanzioni previste da 1.000 ai 4.000 euro in caso di mancata denuncia, spero vivamente, signor Vice Ministro, che il Governo trovi il coraggio e il buon senso di semplificare e alleggerire questa disposizione con il decreto attuativo. Piuttosto di aggravare la burocrazia, in questo caso si dovrebbe pensare - come si fa anche in altre parti d'Europa - a valorizzare e supportare l'apicoltura amatoriale

realtà, a noi basterebbe il limite di 20. Ci sono anche ancora margini importanti per la valorizzazione della qualità dei prodotti. L'agricoltura non può inseguire la logica del prezzo più basso, ma quella della maggiore qualità dei nostri prodotti e delle produzioni d'eccellenza (e noi ne abbiamo in abbondanza). In questo quadro, un contributo molto importante può essere dato dalle giovani generazioni. Il provvedimento contiene un forte impulso in tal senso, che giudico molto positivamente: è un passo nella giusta che ne seguano altri. I giovani possono portare nelle campagne competenze, non solo di carattere tecnico, che sono in grado di mettere a valore la nostra agricoltura anche per i suoi risvolti culturali e sociali, con l'affermazione di valori legati alla qualità della vita. L'Europa, signor Vice Ministro, è un tema a sé. Dall'Europa i nostri agricoltori si aspettano meno burocrazia e più trasparenza. C'è preoccupazione per il TTIP. Le ultime ricerche stimano che - se i termini dell'accordo non dovessero cambiare - il contributo dell'agricoltura al PIL europeo porterebbe ad una diminuzione dello 0,8 per cento, con conseguente perdita di posti di lavoro, mentre quello statunitense aumenterebbe dell'1,9 per cento: una vera e propria ristrutturazione del mercato, che avrebbe effetti anche sulla gestione del territorio e sulle caratteristiche del tessuto produttivo agricolo europeo e italiano. Dobbiamo andarci molto cauti! C'è infine la questione delle quote latte. Il colpo per i nostri allevatori è stato molto forte. Per questo è molto positivo il lavoro che stanno facendo il Ministro e il suo Ministero, cercando di dare un sostegno anche tramite aiuti ed iniziative dirette allo scopo di non fare chiudere altre stalle agli allevatori, soprattutto nelle zone montane e svantaggiate, dove oggi il costo di produzione supera di gran lunga il ricavo per litro. Sono solo alcuni esempi per dare l'idea della vastità e della complessità delle questioni che non possono essere risolte con un singolo provvedimento, occorrendo una forte iniziativa affinché l'agricoltura venga messa al centro dell'agenda politica e istituzionale. L'agricoltura è infatti strategica per il rilancio complessivo del Paese

cui è stata conferita delega, produca norme semplici che vadano concretamente incontro alle esigenze del settore, semplifichino la burocrazia e tutelino soprattutto i piccoli produttori. Signor Vice Ministro, vediamo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto e, con la stessa fiducia che ho espresso nelle premesse, dichiaro il voto favorevole del Gruppo per le

di legge che ci apprestiamo ad approvare rappresenta un tassello importante in un percorso di grande attenzione che il Governo e questo Parlamento hanno dedicato all'agricoltura.

milioni di imprese, il 9 per cento del PIL italiano, tre milioni di lavoratori nella filiera, che rappresentano il 14 per cento degli occupati italiani, e più di 25 miliardi di euro di imposte. Al tempo stesso, è necessario ricordare anche un aspetto negativo e preoccupante: il numero delle nostre aziende agricole si è infatti ridotto dai circa 4 milioni degli anni Sessanta a 1,5 milioni nel 2012. Si tratta di un fenomeno che si è intensificato negli ultimi decenni: dal 1990 al 2000 il comparto ha infatti perso oltre 400.000 aziende e nel decennio successivo ben 775.000. Con l'approvazione del provvedimento in esame si conclude un processo iniziato con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in cui non solo si erano valorizzati strumenti di sostegno alle imprese agricole, ma erano anche state introdotte misure sulla tracciabilità del prodotto agricolo e sulla correttezza e regolarità delle stesse imprese. Nell'ultima legge di stabilità è stato compiuto uno sforzo straordinario per dare prospettiva e strumenti ad un settore che - credo si possa dire senza tema di smentita - rappresenta una delle ossature importanti dei territori del nostro Paese. agricoltura vuol dire, in moltissimi casi, manutenzione del territorio, infrastruttura di base per il turismo, commercio in tante aree marginali del Paese e sostegno a un'economia diffusa e importante. Noi abbiamo lavorato proprio con questa convinzione, cioè che lavorando per l'agricoltura lavoravamo per tutto il Paese. Nel disegno di legge in esame abbiamo inserito misure di semplificazione e provvedimenti importanti per i giovani e le nuove imprese agricole che si insediano. A questo riguardo, credo sia opportuno ricordare che gli interventi che ci apprestiamo a varare sono importanti anche perché, in qualche misura, coincidono con il varo dei nuovi programmi di sviluppo rurale portati avanti dalle Regioni, che dovranno affrontare proprio il tema dell'insediamento dei giovani e la prospettiva delle aziende in tanti territori. Abbiamo affrontato temi riguardanti filiere che possono avere prospettive di sviluppo o che avevano problemi da affrontare e abbiamo poi affrontato aspetti normativi per quel che riguarda l'acquacoltura, la pesca e l'ampio tema del bracconaggio. Sul tema della sburocratizzazione abbiamo approvato misure di semplificazione nell'ambito dell'olio d'oliva, delle denominazioni di origine, della definizione di imprenditore agricolo, in materia di servitù, in materia di riduzione dei tempi per i provvedimenti amministrativi. Ci si è resi conto che è necessario reimpostare complessivamente la struttura legislativa del comparto, che soffre di troppa dispersione di norme e di troppa complicazione nell'applicarle. Dai dati forniti dai sindacati si rileva che un'azienda agricola italiana, per assolvere a tutti gli adempimenti burocratici imposti, spende in media 2 euro ogni ora di lavoro, 20 euro al giorno, 600 euro al mese, 7.200 euro l'anno. All'imprenditore agricolo occorrono otto giorni al mese per riempire le carte richieste dalle amministrazioni centrali e locali. diamo mandato al Governo per una revisione organica della normativa entro tempi precisi, per stilare un codice agricolo che armonizzi i diversi livelli normativi. Peraltro, giova ricordare che con il Piano Agricoltura 2.0 si è anticipato questo obiettivo, introducendo, attraverso un avanzato sistema informatico, la semplificazione dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i comparti dell'agricoltura e della pesca. Nel piano sono contenute le domande precompilate, un'unica banca dati certificata e l'anagrafe unica delle aziende. Gli adempimenti che gli agricoltori dovevano compilare separatamente si semplificano e si sintetizzano in un unico fascicolo aziendale. Sono interventi di buonsenso, che non solo tendono alla semplificazione burocratica, ma che intendono valorizzare piccole realtà, spesso presidi preziosi dei territori più marginali. Sotto questo aspetto, assumono grande importanza i nuovi strumenti per favorire i processi di affiancamento economico e gestionale di giovani nell'attività di impresa agricola. I dati sull'occupazione dei nostri giovani registrano infatti un crescente interesse per il ritorno alla terra. In qualche misura, sono semplificazioni importanti anche l'aver affrontato la riforma del quadro normativo della silvicoltura, quanto mai necessaria,

che hanno avuto l'ambizione di prendere in mano proprio il tema della semplificazione, provando a coniugarlo in modo concreto e puntuale, laddove c'erano questioni che chiedevano di essere affrontate. Per quanto riguarda i giovani, abbiamo inserito in questo provvedimento una norma sulle società di affiancamento e sulla banca della terra. Si tratta di misure importanti, proprio perché hanno l'ambizione di accompagnare quel processo in atto, sostenuto soprattutto con i programmi di sviluppo rurale e di reinsediamento, e di garantire una prospettiva a quelle a quelle aziende che naturalmente non ce l'avrebbero. Credo che parlare di questi temi voglia dire parlare di gran parte dei territori appenninici della nostra Italia, ma anche di fette importanti di aree pedemontane e collinari svantaggiate; un tema assolutamente fondamentale. Altro aspetto toccato dal collegato è quello della riorganizzazione di enti, a partire dal campo dell'assistenza tecnica in zootecnia e degli enti vigilati e partecipati dal Ministero. Così come importante è la delega per la riforma del settore ittico, che richiede veramente un intervento urgente, proprio perché è un *asset* rilevante. Abbiamo affrontato questioni inerenti al pomodoro e al riso. Voglio solo citare la delega al riso, importante anche perché nasce da una condivisione globale di tutta la filiera su come regolamentare, alla luce delle nuove necessità, il tema della valorizzazione e della commercializzazione di questo prodotto. Abbiamo affrontato il tema dell'apicoltura e quello della birra artigianale, un piccolo settore, ma fiore all'occhiello delle nostre produzioni tipiche di qualità del territorio. Per il settore della birra si sono introdotte norme a tutela dei piccoli birrifici con produzione inferiore ai 200.000 ettolitri, che daranno grande slancio ad una produzione artigianale molto spesso portata avanti da giovani imprenditori; un fenomeno straordinario, che in pochi anni è cresciuto in modo importantissimo. Credo che ormai siamo prossimi ai mille birrifici artigianali, coprendo una quota pari quasi al 3 per cento del consumo di birra nel nostro Paese, che rappresentano quantitativamente numeri non comparabili con gli impianti industriali, ma che sicuramente rappresentano la punta di diamante di una qualità italiana che sta conquistando, anche all'estero, riconoscimenti e apprezzamenti per la qualità e l'innovazione che ha saputo mettere in campo. come è già stato detto, era prevista nella versione originale di questo provvedimento una serie di norme in tema di acquacoltura e pesca; si è deciso di lasciar fuori gran parte di tale normativa proprio perché alla Camera dei deputati sta emergendo un testo organico su questa materia. Si è però deciso di mantenere nel provvedimento in esame il tema delle sanzioni, proprio perché è a sé stante e necessitava di essere trattato. È stato poi introdotto nel dibattito in Commissione alla Camera il tema del contrasto al bracconaggio, un passo importante in termini di civiltà giuridica e di rispetto degli animali, dell'ambiente e di chi sul territorio ha l'ambizione di vivere rispettando le regole. regole. Un'ultima annotazione. Uno degli articoli finali del provvedimento riguarda una definizione puntuale dei materiali che vengono utilizzati per il biogas, che non vengono più definiti come rifiuti. Può sembrare una piccola cosa, è un piccolo articolo; ma per chi ha lavorato sui territori si tratta di una norma che risolve diversità di interpretazione da territorio a territorio, situazioni complesse che si vengono a creare su questi temi: con un'interpretazione univoca che credo si potrà dare prospettiva ad un settore, quello del biogas, che contiene in sé la potenzialità di produrre energie valorizzando materiale che comunque degraderebbe di suo nell'ambiente, e che merita quindi questo tipo di valorizzazione. Penso di poter dire che il lavoro fatto sia stato assolutamente importante. Lo è per l'agricoltura, che in questa stagione sta sicuramente attraversando una fase molto complessa, ma che al tempo stesso sta esprimendo delle potenzialità straordinarie, soprattutto per quel che riguarda l'*export* dei prodotti di qualità. Superiamo abbondantemente i 37 miliardi di euro di prodotto esportato, e l'orizzonte che ci si era definito, dei 50 miliardi nel 2020, non non è più così lontano. Come ho detto all'inizio del mio intervento, parlare di agricoltura vuol dire parlare di ciò che riguarda la vita di tanta parte dei nostri territori: in questo senso la soddisfazione che proviamo è grande, perché abbiamo lavorato per l'agricoltura, ma attraverso essa abbiamo lavorato per tutto ciò che c'è di grande, di potenzialmente importante per l'economia e il futuro dei territori. Un'ultimissima considerazione. Voglio esprimere tutto l'apprezzamento per come si è svolto il lavoro in entrambi i rami del Parlamento e ringraziare tutti i Gruppi che hanno contribuito a questo lavoro, perché è stato veramente un grande gioco di squadra. Ringrazio il presidente Formigoni, la Commissione

sono trascorsi più di due anni ormai dal lontano 21 febbraio 2014, data in cui questo provvedimento è approdato per la prima volta in Senato. è diventato una barcaccia, o meglio lo scafo dei peggiori traghettatori con a capo il vostro scafista specializzato in marchette preelettorali e postelettorali. Un testo che ormai si riassume, tra le altre, nelle solite deleghe al Governo. Infatti, si traghettano disposizioni in materia di contratti agrari, si tratta la parità tra ì sessi nei consorzi di tutela

Niente più semplificazione e razionalizzazione né tantomeno competitività, quindi nessuna misura adeguata per il comparto agricolo ma, al contrario, tutto è stato concesso per favorire le *lobbies* ed i poteri più o meno occulti che il signor bancarotta ha dovuto accontentare per la gioia di "Santa Maria Etruria". Cominciamo con l'articolo 1 - e direi che già cominciamo male - perché il comma 10 viene a modificare una disposizione del decreto-legge competitività che di competitivo non aveva nulla - ed aggiunge agli ambiti operativi del sistema di consulenza anche gli aspetti che riguardano: l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario. Noi riteniamo che questa ultima definizione sia troppo generica e potrebbe costituire una pericolosa apertura alla coltivazione di OGM. Per questo motivo abbiamo chiesto: o di sopprimere il riferimento a questo ambito oppure di precisarlo o circoscriverlo. Ma niente. Nulla di tutto questo è stato concesso. Questo, ovviamente, evidenzia la vostra chiara intenzione, quella di aprire alle coltivazioni OGM. pesca e acquacoltura, chiediamo la reintroduzione di specifici criteri di delega, perché il riordino e la semplificazione deve riguardare anche questo settore, che non bisogna lasciare nel dimenticatoio. Inoltre, in ogni caso, una delega al Governo non può e non deve essere la solita carta bianca dove scrivere quello che si vuole. Le Commissioni competenti devono rendere pareri obbligatori e vincolanti, senza i quali i Dicasteri interessati non possono fare niente. Abbiamo chiesto che dall'attuazione delle disposizioni sull'affiancamento per le terre agricole non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È assurdo ancora caricare i contribuenti di spese che, unite ad altre, diventano sempre più insostenibili. Quindi, non parlate di ripresa e di riforma, ripresa e di riforma, perché non avete fatto altro che affossare il comparto. All'articolo 8, abbiamo proposto di aiutare gli imprenditori dei territori montani o svantaggiati in riferimento alla disciplina delle attività affidate in subappalto. Ma niente: anche questo è stato respinto. la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi diritto alle indennità espropriative giacenti, deve essere a titolo gratuito, così come l'accesso alle banche dati nazionali dell'anagrafe zootecnica per i produttori di latte nell'ambito dei piani di sviluppo rurale. Infine, sempre a proposito di denaro, abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo 10 riguardante il contributo al CONOE. Proseguendo, e in tema di trasparenza, l'attività di manutenzione del verde deve essere esercitata attraverso procedure di affidamento trasparenti, con un bando ad evidenza pubblica, privilegiando imprese che usano metodologie a basso impatto ambientale. Non è sufficiente la sola iscrizione al registro ufficiale dei produttori. Ma anche su questo, niente. inoltre proposto che il sistema di tracciabilità del riso diventi obbligatorio; che le disposizioni in materia di prodotti derivati si applichino anche al pomodoro coltivato e trasformato in Italia, con etichette chiare non solo per il miele, ma anche per i prodotti apistici.

Ed è proprio il caso di dire: ma datevi all'ippica che forse fate meno danni. Riformare e rilanciare un settore vuol dire, prima di tutto, utilizzare gli strumenti normativi più adeguati. E invece no:

non si può tralasciare che l'organismo pubblico-privato ippico ha dei compiti assai delicati, che vanno dall'organizzazione di eventi ippici alla ripartizione e rendicontazione delle risorse. quindi, non basta - come impropriamente fa il testo del collegato - che la disciplina degli organi di governo sia improntata a criteri vaghi, a qualcosa che non è scritto e che poi va interpretato, come i criteri di rappresentanza. Per questo abbiamo chiesto che l'organismo faccia riferimento anche ai soliti nostri criteri di trasparenza e pubblicità. Un aspetto su cui tra l'altro la Commissione europea aveva già fatto dei rilievi, proprio sul rispetto dei principi di libera prestazione dei servizi, di libertà di stabilimento e di trasparenza. La massima divulgazione delle informazioni è alla base, non solo di una cittadinanza attiva, ma anche di una società democratica ed evoluta. Il pericolo, poi, che i componenti, specie ministeriali, dell'organismo ippico possano avere dei conflitti di interesse rispetto alle cariche che rivestono è reale. Per questo siamo intervenuti con un emendamento per eliminare qualsiasi effetto distorsivo. Ma voi volete continuare a distorcere. restando sempre in tema ippico, si liquidano con soluzioni normative improprie questioni che avrebbero bisogno di un approccio più pragmatico, rispetto al quale avete dimostrato, ancora una volta, di essere totalmente incompetenti. Non basta autodelegarsi come vergognosamente continuate a fare. Le questioni non si risolvono a colpi di accetta. Abbiamo chiesto l'inasprimento delle disposizioni riguardanti il contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne, sia con sanzioni più severe, sia vietando pratiche nemiche degli equilibri faunistici, come ad esempio l'utilizzo di reti, attrezzi e strumenti difformi. Ma non basta, perché, *dulcis in fundo*, ci sono sfalci e potature. ci permettiamo di fare un'equazione, perché con il passaggio alla Camera è saltato fuori un articolo che sta all'agricoltura come il Governo sta al buonsenso; cioè, tanto per rimanere in tema agricolo, un fico secco. Si tratta, nello specifico, di una modifica all'articolo 185 del codice ambientale, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti; un altro frutto amaro dell'albero delle magiche trovate del PD. per farla breve, dentro un collegato agricolo vi siete inventati di manipolare il codice ambientale - di palo in frasca, sempre per rimanere in tema agricolo - e avete deciso di escludere dalla definizione di rifiuto le materie fecali, la paglia, gli sfalci, le potature e compagnia cantando. Questo è un punto, tra l'altro, già evidenziato dalla relazione del servizio di bilancio del febbraio di quest'anno. Allora diteci: se non lo considerate un rifiuto come lo considerate? Ma soprattutto: come pensate di eliminarlo? E qui si apre un mondo, perché l'eliminazione di questi rifiuti potrebbe generare degli incenerimenti. Dove? Come?

provate invece a bruciare i tempi e magari a restituire i rimborsi del versato dell'IMU agricola degli anni 2014 e 2015. Bruciate questi di anni, anziché altro. L'agricoltura ancora una volta fa la Cenerentola dei tre comparti economici, un settore che prima strumentalizzate per Expo e che poi massacrate anziché provvedere a legiferare con buonsenso per questo settore.

non può avere il nostro voto favorevole e nemmeno il nostro voto contrario, per cui annuncio il nostro voto di astensione. Concludo dicendo ancora una volta che non servono le deleghe, non servono arbitri o squadre che poi si vendono al migliore offerente. Questo delegato è solo l'esempio della strage normativa che state facendo, perché i vostri provvedimenti hanno un unico padrone: il mercato dei pasticci. Un provvedimento, per finire, che ha coinvolto quattro elementi naturali: terra, aria, acqua e purtroppo pure il fuoco. Fuoco sparato sopra a colpi di lanciafiamme e che impedisce, di fatto, di poterci esprimere positivamente. Perché da questo collegato si evince solo una cosa: volete la delega per far arrivare il latte dalla Romania, importare pomodori dalla Cina, l'olio dalla Tunisia, grano dal Mar Nero, *stock* ittici dal Pacifico. E di italiano cosa rimane? La vostra riforma su questa schifezza e la vostra firma su questo collegato agricolo.

come è già stato sottolineato da qualche mio collega giunge oggi alla definitiva approvazione, dopo oltre ventisette mesi dall'avvio del suo esame, il collegato agricolo alla manovra di finanza pubblica del 2013. Un provvedimento che è stato presentato dal precedente Governo (quello a guida Letta, per intenderci) e che è stato oggetto di vari e importanti rimaneggiamenti, come l'ultimo avvenuto alla Camera,

è intervenuta nuovamente la Camera, che ne ha sostanzialmente abolito ogni elemento di arricchimento costringendoci oggi a prendere atto del suo lavoro senza possibilità di intervenire. Sulla base di questa metodologia, nonostante il tempo e il lavoro parlamentare profuso su questa iniziativa (forse un tempo troppo lungo), resta evidente la presenza di tare, che limitano quelle che erano le potenzialità di un provvedimento coraggioso e incoraggiante per l'intero settore; un provvedimento che tutti auspicavano fosse organico e che avesse l'ambizione di rilanciare. Da questo punto di vista, credo sia stato un peccato che sia mancata l'ambizione e la forza necessarie a questo impegno dal punto di vista politico, in un progetto che comprendevo e comprendo benissimo essere arduo, ma che, allo stesso tempo, consideravo e considero stringente e necessario. Così, alcuni buoni propositi, penso si sia perduta un'altra occasione. Penso che si sia perduta un'altra occasione quando l'introduzione dell'articolo 9 e dell'articolo 15 venir meno la possibilità di essere realmente incisivi sullo stato dei luoghi. Ma è stata anche un'opportunità perduta, credo, la scelta di una serie di provvedimenti e disposizioni, che si sono sviluppati in maniera parallela e autonoma, ma che comunque afferivano alla materia del presente provvedimento, che sono transitati con altre iniziative legislative, svilendo in parte o in gran parte - proprio l'intendimento principale di questo provvedimento, che era quello di essere organico, di costituire una piattaforma complessiva del sistema agricolo, per provare a risolvere alcuni elementi di difficoltà, soprattutto in termini di semplificazione.

hanno rafforzato - se così posso dire - la timidezza insita nel disegno di legge iniziale. Come se non bastasse, tutte queste iniziative parallele non sempre hanno segnato un reale vantaggio per questo settore, come, ad esempio e da ultimo, il parere favorevole dell'Esecutivo alla mancata indicazione della scadenza dell'olio di oliva. Sia ben chiaro: non mi illudevo, né pensavo fosse possibile la redazione di un vero e proprio Zibaldone sull'agricoltura e per l'agricoltura. però, se parliamo di razionalizzazione e semplificazione, come riportato in titolo a questo disegno di legge, continuare a vedere la frammentazione di questa materia in diversi rivoli e provvedimenti non rende particolarmente facile, né concreto immaginare di poter raggiungere l'obiettivo. È questo motivo che mi spinge - e che ci spinge - a considerare questo provvedimento un'occasione perduta, almeno in grandissima parte, e che ci spinge ad operare nella direzione di un voto di astensione sul

risolta, perché così noi rischieremo di non essere in grado di dare risposte efficaci, o perlomeno di dare quelle risposte a un settore tanto strategico quanto capace di tener testa più di altri alla crisi e che ripone particolare fiducia in un provvedimento che avrebbe dovuto aggredire lacci e lacciuoli che ne strozzano il rilancio complessivo. che manchi ancora chiarezza e univocità nella linea da perseguire in questo campo a partire - lo ribadisco anche oggi - da quella da tenere in Europa, dove dobbiamo condurre la madre di tutte le battaglie, cioè quella volta a preservare la produzione italiana e la sua qualità, ad opporci a provvedimenti che vogliono standardizzare le produzioni di tutti i Paesi europei, quella diretta a combattere la concorrenza sleale e ad adoperarsi per una efficace tutela del territorio e quindi anche delle sue identità e produzioni. Le ricadute positive di Expo rischiano di non raggiungere l'auspicato medio periodo senza una strategia effettiva che combini la semplificazione con l'innovazione,

confermo il voto di astensione da parte mia personale e del Gruppo; un voto di astensione che è l'ennesimo atto di di riconoscimento di una volontà alla quale non ha corrisposto un lavoro al quale non ci siamo sottratti, perché anche in Commissione l'impegno è stato importante; lo dico rivolgendomi

forse gli è stata consegnata) di esprimere parere favorevole a qualsiasi iniziativa di miglioramento. Eravamo consapevoli che il tempo trascorso fosse tanto, ma eravamo altrettanto fiduciosi che i suggerimenti che potevano migliorare l'efficacia del provvedimento forse voleva la pena fossero raccolti. Confermo quindi il nostro voto di astensione. Signora Presidente, onorevoli colleghi, agricoltori che da casa ci ascoltate e ci guardate, credo anche stupiti da quante cose sono state dette oggi. Mi riferisco in particolare a questo

mi avrebbe fatto piacere avere anche il Ministro in questa sede oggi, ma purtroppo è una figura che non ci degna della sua presenza e mi dispiace profondamente che il Ministro delle politiche

veramente potrebbe trasformarlo e tradurlo in qualche articolo di legge. Dicevo se vi siete mai presi la briga di andare a vedere qual è il reddito medio dell'agricoltore italiano. Siete mai andati a vedere il livello di spesa parametrato al reddito dell'agricoltore? Se andaste a vedere, probabilmente vi rendereste conto che l'opinione per cui l'agricoltura oggi fiorisce in un modo esagerato

per cento. Andate a vedere quanto è aumentato il reddito degli agricoltori italiani. Si fa riferimento a dati Eurostat, presumo del 2015. Ma andate a vedere quelli del 2014, il reddito degli agricoltori era calato dell'11 per cento. Facciamo un discorso a livello generale e finiamola di prendere in giro gli agricoltori dicendo che l'agricoltura va bene. Oggi, chiedetevi cosa

qui si vuole apparecchiare la tavola e si studia come apparecchiarla correttamente quando il cibo non c'è. C'è un metodo decisamente sbagliato nell'affrontare i problemi dell'agricoltura.

dell'attribuzione del diritto di prelazione a favore dell'imprenditore agricolo professionale rispetto ad altre figure. Mi chiedo cosa avete inventato di nuovo. È qualcosa che già c'era nel diritto di prelazione di chi è confinante. Non sarà mica un'innovazione!

è stato soppresso l'articolo che prevede la modernizzazione della logistica. Vorrei mi si spiegasse il perché di questa

Si è parlato di agricoltura sociale, biodiversità, legge di diversificazione, quasi fossero medaglie da apporre al petto di questo Governo. Sono però disposto a confrontarmi e a sfidare il Governo in qualsiasi momento,

di politica agricola che, sin dal suo insediamento, il Governo Renzi e la maggioranza parlamentare hanno indicato per superare le fragilità strutturali del sistema produttivo: l'inefficienza e l'inefficacia degli strumenti pubblici di supporto, l'inadeguatezza del sistema di gestione dei rischi, il fenomeno di sfruttamento del lavoro, nonché le storture di una concorrenza spesso sleale. È però innegabile

e di tracciabilità, riavvicinando i consumatori a produttori non più anonimi e indistinti. Si sono affermate inedite modalità di ricomposizione di un reddito, assottigliato da logiche di un mercato sempre più difficile e complesso, che ha progressivamente ridotto i prezzi e richiesto maggiori *performance*. Questo va loro riconosciuto. Queste imprese, che oggi sono una minoranza distribuita a macchia di leopardo sul territorio nazionale, rappresentano però il prototipo di un nuovo modello. Sono imprese che hanno saputo costruire una loro forza competitiva, basata su ricerca e investimento in qualità e salubrità del prodotto, rafforzata da tanti elementi immateriali (il modo di produrre, il legame con i luoghi, le conoscenze, la capacità di mettere insieme e ottimizzare tradizione e innovazione), incrociando aspettative sempre più sofisticate di una domanda consapevole e competente. Con loro abbiamo parlato e ci siamo confrontati sui nodi strutturali, in una quotidianità che ha continuato a essere fatta di calamità naturali, di fluttuazioni dei prezzi, di crisi di settori importanti: dal lattiero-caseario all'olivicolo, dal suinicolo al cerealicolo, al bieticolo-saccarifero, dalla pesca all'acquacoltura, solo per ricordare i principali. Abbiamo puntato con decisione su un nuovo protagonismo delle imprese, sul ricambio generazionale, sull'aggregazione dell'offerta e l'integrazione tra imprese nelle filiere, sull'innovazione degli strumenti della gestione - sempre più complessa - del rischio e dell'accesso al credito. Stiamo perseguendo trasparenza nella tracciabilità e abbiamo lanciato una sfida multilaterale vera verso la legalità. Questi sono gli assi di un lavoro parlamentare che dovrebbe inorgoglirci tutti e che nella legislatura precedente voglio ricordarlo - ha sempre trovato Governi sordi, Ministri precari, assenza di indirizzi, mancanza di rapporti con l'Unione europea. L'accelerazione data dal Governo Renzi a intervenire, ammodernando e innovando, i settori agricolo e agroalimentare ha aperto, di fatto, una nuova stagione legislativa, proprio partendo dal testo del collegato. Cari amici, per me sono stati due anni straordinari, assolutamente eccezionali, per l'agricoltura, l'agroalimentare, la pesca e l'acquacoltura. anche per il nostro impegno e la produttività del nostro lavoro qui, al Senato; un impegno di tutti quanti, all'interno della 9a Commissione, nel confronto con il Governo, con il Ministero, con la Camera, ognuno nel nel proprio ruolo. Sicuramente ci abbiamo messo tanta passione e tanto spirito di rappresentanza dei nostri territori, anche da parte di colleghi impegnati in altre materie. materie. Il vento è cambiato. Il nostro lavoro ha veramente inciso sulle scelte che stanno accompagnando la trasformazione di questi settori, con una nuova centralità nella politica economica, sociale e ambientale del Paese. Sono state affrontate le cause dell'arretratezza; si è ricostruito un nuovo rapporto tra produttore e consumatore, trovando come chiave di volta un potenziale straordinario, fatto di prodotti di qualità, di agricolture rispettose dell'ambiente, di lavoro dignitoso ed equamente retribuito.

tralasciando l'interesse ad assumerci la paternità delle nuove proposte a favore dell'obiettivo della loro concretizzazione. Campo libero nel cosiddetto decreto competitività; decreti d'urgenza per i settori del latte e dell'olio e in tema di calamità naturali; agricoltura sociale; biodiversità; riduzione del carico fiscale con l'esenzione IMU e IRAP per le imprese agricole; contrasto allo sfruttamento del lavoro; testo unico sul vino; consumo del suolo; ristorazione collettiva; educazione al valore del cibo; settore della canapa; testo unico sulla pesca e sull'acquacoltura (e non una delega);

Molte parti sono state stralciate, ma non sono sparite in quanto confluite in altri provvedimenti (come, ad esempio, per la pesca e l'acquacoltura), così come i nuovi inserimenti alla Camera dei deputati da nuovi argomenti portati alla nostra attenzione (mi riferisco, ad esempio, alla birra artigianale e al settore apistico). Cari colleghi, credo che porterò il provvedimento che mostra tutta l'inefficienza del bicameralismo paritario, come esempio per sostenere il sì al *referendum* sulla riforma costituzionale. Expo è stata un'occasione straordinaria di lancio internazionale del *brand made in Italy*, dietro al quale vi sono valore vero, unicità, sicurezza e salute. Si è trattato di un pezzo importante della nostra battaglia contro l'*italian sounding*, che non si fa pensando solo a barriere. Sicuramente abbiamo bisogno di rafforzare, come già abbiamo fatto, i controlli contro la contraffazione, ma per proteggere i nostri *brand* all'estero dobbiamo lavorare e collaborare con i Paesi che più mostrano interesse per i nostri prodotti. però non è stato solo questo. Dalle politiche di settore sono usciti messaggi per tutti sul valore del cibo e un'assunzione di responsabilità ad affermare nel mondo il diritto universale al cibo come obiettivo per nuove politiche di uguaglianza e lotta alle disuguaglianze. La centralità dell'agricoltura apre nuove opportunità, ma anche nuove sfide sulle quali abbiamo solo iniziato a discutere e per le quali sono molto lontane sintesi condivise. Quale rapporto tra scienza e politica, tra scienza e produzione, tra nuove tecnologie e futuro delle produzioni? Quali relazioni commerciali con gli altri Paesi? Il lavoro da fare è sicuramente ancora tanto. Alcune consegne sono già contenute nel provvedimento sulle stesse deleghe che stiamo dando al Governo e su cui ci sono forti aspettative, anzitutto con riguardo alla semplificazione normativa. Questo Paese non è mai riuscito a dotarsi di un codice agricolo

superiore al risultato ottenuto negli altri settori economici del nostro Paese. Ma il dato più eclatante è che per la prima volta i dati di crescita delle Regioni del Sud sono più alti della media nazionale. Aumenta l'occupazione nel settore, come pure aumenta la resa produttiva e il margine di reddito. Quest'ultimo dato, relativo alle Regioni del Sud, è senz'altro il risultato più significativo, perché si riferisce ad un settore che là tradizionalmente viene marginalizzato in termini di competitività, sia perché viene da quella parte del Paese che più faticosamente stenta a ripartire. È vero, si tratta di un dato statistico e, come tale, ha bisogno di essere scomposto e meglio approfondito,

che sia anche il frutto delle politiche di riforma e di investimento di questo Governo e di questa maggioranza. Ciò non sta avvenendo per circostanze casuali e non è neppure temporaneo. È frutto di un processo di cambiamento vero nel ruolo che la produzione di beni primari sta subendo, in una società che si trasforma e con un rinnovato rapporto con il cibo, con la salute e con l'ambiente, e di una politica che lo sta intercettando, sostenendo e rafforzando. Andiamo avanti su questa strada, il PD ci sarà convintamente.

particolarmente significativo per la complessità delle questioni che si dovevano affrontare e soprattutto per la necessità di un punto di equilibrio tra esigenze opposte ed entrambe meritevoli di grande considerazione. Quindi, si tratta di un caso nel quale il legislatore deve essere dotato di quella capacità di equilibrio che deve comportare una norma che sia poi fruibile per l'autorità giudiziaria, la quale sarà chiamata ad applicarla. Primo punto. Si tratta, nella sua ipotesi base, di un delitto comune, ossia di un delitto che può essere commesso da ogni cittadino. La Commissione, infatti, ha inteso determinare una tutela ancora più rafforzata che non nel caso in cui il reato fosse stato costruito esclusivamente sulla figura del pubblico ufficiale. La tutela è più rafforzata perché chiaramente amplifica il campo di applicazione della norma, rendendola ovviamente applicabile ad ogni contesto, quindi anche a quello non pubblicisticamente qualificato. In che cosa consiste la struttura del fatto? Nel testo, perlomeno quello giunto al Senato, si parla di violenze, minacce gravi e reiterate, ovvero di avere agito con crudeltà nei confronti delle vittime; che abbiano determinato una condizione di acute sofferenze fisiche a carico della medesime persona offesa,

Ma, queste acute sofferenze fisiche o questo verificabile trauma psichico devono essere compiuti nei confronti di un soggetto privato della libertà personale. Onorevoli senatrici e senatori, questa scelta è stata in un certo senso dettata dalla necessità di differenziare - è un punto penalisticamente molto delicato - questo reato dalle pur contestabili, a prescindere dall'introduzione dall'introduzione di questa norma penale incriminatrice, norme di riferimento. Infatti, una delle difficoltà nello scrivere e nel pensare al delitto

è chiaro che già commette un reato a prescindere dall'introduzione del delitto di tortura. Questo lo dico perché è chiaro che questa condotta andava seriamente diversificata, altrimenti non si sarebbe compreso il perché di una criminalizzazione di condotte precedentemente criminalizzate. La figura del pubblico ufficiale è stata invece prevista, perché andava fatta, nell'ipotesi aggravata, con una disposizione che sostanzialmente rinvia alla struttura base del fatto, perché si limita a dire che se il fatto di cui al comma precedente è compiuto da un pubblico ufficiale ovviamente le pene sono aggravate. Ma qui non si introduce nessun elemento ulteriore di fattispecie se non l'indicazione

all'interno dello stesso articolo 1 che contempla il delitto di tortura, l'istigazione alla tortura. Si tratta anche qui di un reato di istigazione che sancisce un'eccezione a principi storici del diritto penale, ma che qui si comprende per la gravità dei fatti, ancorché si tratti di una istigazione particolare: quella del pubblico ufficiale nei confronti del pubblico ufficiale e dell'istigazione dell'incaricato di un pubblico servizio nei confronti di un soggetto analogo. Quindi, è una istigazione che avviene in un ambiente chiuso, in determinati contesti, avendo ritenuto la Commissione di considerare questi fatti particolarmente gravi. Ragionando in senso opposto rispetto a una certa tradizione in materia di istigazione, si è ritenuto che una istigazione limitata a un determinato contesto, contesto, caratterizzato dalla presenza di più persone, potesse avere una maggiore diffusività. Concluderei qui il mio intervento, avendo dato delle indicazioni soltanto sommarie sulla struttura del delitto di tortura. Poi, il disegno di legge si compone ovviamente di altre disposizioni, delle quali parleremo variamente nel corso dei lavori parlamentari. Si stabilisce, per fare delle semplificazioni, che le prove ottenute attraverso tortura (qui si pensa, ovviamente, a contesti investigativi) sono inutilizzabili. È una norma necessaria, ancorché la giurisprudenza, ma anche la dottrina, abbiano da sempre elaborato la categoria delle prove illecite. È fuor di dubbio che se la prova è frutto di un'attività violenta la prova sia inutilizzabile. Si stabilisce che non possa essere riconosciuta alcuna immunità ad agenti, anche militari, di Governo stranieri che siano indagati o già condannati per il delitto di tortura. a corredo di questa norma generalista sulla tortura, si dicono tante cose, tra le quali anche, conclusivamente, l'affermazione secondo la quale non sono consentiti espulsioni e respingimenti ovvero la estradizione nei confronti di una persona rispetto alla quale vi sia il concreto pericolo che, se restituita al Paese d'origine, sarebbe sottoposta a tortura, tenendo conto anche, nel contesto di un simile giudizio, della sistematica violazione dei diritti umani nel Paese dove quel soggetto dovrebbe ritornare.

Signor Presidente, senatrici e senatori, signor rappresentante del Governo, ritengo questa discussione tanto importante quanto delicata. Voglio ricordare che questo disegno di legge prevede l'introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie penale del delitto di tortura,

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura è del 1984. La ratifica da parte del nostro Paese è del 1988. Sono appunto Voglio ricordare che il 15 marzo 2013 ho presentato un disegno di legge sul delitto di tortura, sottoscritto anche dai senatori Corsini e Tronti, che faceva puntuale riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite e al suo principio ispiratore. Il testo che oggi stiamo discutendo, a mio avviso, è assai lontano da quella che era l'ispirazione della Convenzione internazionale, innanzitutto per un motivo che va evidenziato e per una ragione assai significativa. In altri ordinamenti e nel disegno di legge da me e da altri presentato, il reato di tortura viene definito come reato proprio, attribuibile cioè ai pubblici ufficiali o a chi esercita pubblico servizio. In questo non c'è alcuna forma di accanimento contro le forze di polizia o tantomeno un preconcetto, una sorta di ostilità nei confronti degli apparati dello Stato, bensì la consapevolezza che la tortura trovi il suo fondamento, la sua ragione d'essere e il suo quadro più pertinente e coerente in una categoria cruciale: l'abuso di potere. La tortura non è in questo contesto un'inclinazione perversa, non è la manifestazione di una psicopatologia individuale, non è l'efferatezza di un singolo. Come giustamente ha rilevato il presidente D'Ascola, per questi comportamenti, per l'esercizio della violenza fisica e psichica tra i privati, il nostro ordinamento prevede fattispecie penali precise e adeguate sanzioni. No, il reato di tortura è qualcosa di molto diverso: è l'esercizio di una violenza fisica o psichica da parte di chi detiene il potere sul corpo di un altro. La tortura è quel comportamento che infligge acute sofferenze, messo in atto da parte di chi ha la titolarità legale della custodia di una persona privata della libertà. Questa è l'essenza fondativa del reato di tortura, sia nella Convenzione internazionale, sia negli ordinamenti di Stati democratici a noi affini. di tutto ciò, rispetto al testo di cui stiamo discutendo, non resta traccia, perché il reato di cui parliamo è diventato un reato comune, ovvero quello che si può commettere nelle relazioni tra i privati. Ma del testo in discussione, che appunto solleva in me robuste perplessità e diffusi dubbi, voglio evidenziare due elementi: il primo è che, rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato, alla formula «violenze fisiche o psichiche» è stato aggiunto il termine «reiterate». Si pensi che in origine la formula è «violenza fisica o psichica», bastando appunto, come dice la Convenzione della Nazioni Unite, «qualsiasi atto» capace di infliggere acute sofferenze perché vi sia tortura. Quel «qualsiasi atto» diventa un plurale («violenze fisiche e psichiche») e a questo plurale si aggiunge un altro termine: «reiterate». Temo che ciò incoraggi una tendenza macabra e causidica, una sorta di numerologia, una fosca aritmetica delle crudeltà che indica una soglia oltre la quale si ha tortura, il «quante volte», e prima della quale non si ha tortura. Ricordo che durante la XIV legislatura, esattamente per questo motivo, il presidente della Commissione giustizia, onorevole Pecorella, chiese e ottenne che il testo venisse rimandato in Commissione, perché, appunto, aveva evidenziato quella tendenza irresistibile verso una vocazione classificatoria che rendeva gli atti di tortura una sorta di sequenza *splatter* di un film *horror*. Non solo: l'originaria formulazione «violenza psichica» è stata sostituita da un'altra: «verificabile trauma psichico». Su questo io ho fatto qualche ricerca, ho avuto numerosi colloqui, ho provato ad indagare e ad approfondire. Vedrete che la letteratura scientifica internazionale sottolinea una circostanza singolare: quella che nella iconografia filmica e letteraria è la più ricorrente delle circostanze di violenza psichica, quella che comunemente viene definita *roulette* russa, secondo la letteratura scientifica internazionale è un comportamento, il cui esito non è tra quelli verificabili clinicamente come un trauma psichico, nonostante esso sia potuto accadere a poche ore di distanza dalla verifica scientifica. Dunque, io ritengo che queste ulteriori specificazioni corrispondano ad altrettanti ostacoli, limiti posti all'accertamento di quell'atto di tortura che, a mio avviso, molto più saggiamente doveva essere affidato alla capacità di discernimento dell'autorità giurisprudenziale. Questo fa sì che il mio atteggiamento nei confronti di questo disegno di legge sia di estrema perplessità e vorrò verificare l'esito

della vicenda di Giulio Regeni. Non ho voluto intervenire, anche perché il solo fatto che quell'atroce vicenda sia ormai diventata, nei nostri archivi della memoria, il caso Regeni mi sembra neutralizzarne la portata drammatica e ridurla, appunto, a una sorta di intollerabile serialità degli accidenti della storia. Ma oggi non voglio aggiungere mie personali considerazioni, fedele alla volontà di sottrarmi a un dibattito che ho considerato spesso superficiale. Voglio, però, ricorrere alle parole

Senato, in questa istituzione, il martedì di Pasqua. Paola Regeni è una donna che, forse in virtù di quella grazia di stato che la teologia cattolica riconosce in chi si trovi in condizioni di estrema sofferenza, sa trovare parole di una potenza letteraria e civile davvero rare. Paola Regeni ha detto: «Ho visto il volto di mio figlio diventato piccolo, piccolo, piccolo. In quel volto ho visto tutto il male del mondo». mondo». La tortura non è semplicemente un atto di crudeltà che colpisce le carni di un individuo; è volontà di annichilimento della persona e volontà di mortificazione e degradazione della sua dignità. È per questo che chiedo

Signor Presidente, forse è qualche anno che stiamo valutando questo disegno di legge e arriviamo qui ancora a modificare, come è stata modificata in Commissione, la proposta che era partita in questa sede, è andata alla Camera e ha avuto un sostanziale mutamento. Forse sono anni che denotano il fatto che su questo tema probabilmente non si è trovato quell'equilibrio di cui parlava il presidente D'Ascola. Non lo si vede quell'equilibrio, perché il testo varato dal Senato in prima lettura poi alla Camera dei deputati è stato completamente modificato in una maniera del tutto incomprensibile e per noi assolutamente inaccettabile. Non possiamo però tacere di questo passaggio che è stato fatto, perché fino a prova contraria, al di là di alcune precisazioni,

che in realtà non si arrivava a punire quel reato di tortura come lo si potrebbe immaginare nel diritto naturale, ma si andava a trovare un insieme di comportamenti per cui alla fine c'erano una certa indeterminatezza e genericità che rischiavano di sfruttare la tipologia di reato al fine di punire condotte che non avevano niente a che vedere con la tortura. Ricordiamo - perché ora non si può tacere - la polemica sorta da parte delle stesse forze di polizia.

*morituri*, in Commissione abbiamo rilevato degli elementi giuridici e cercato di contenere la fattispecie con quell'equilibrio di cui parlava prima il Presidente. Allora dico che probabilmente si parla di equilibrio nella nuova formulazione dell'articolo 613-*bis*

serviva proprio a cercare di contemperare questa configurazione di reato e di distinguerla, o quantomeno serviva a non arrivare a configurarla ogni qualvolta un agente

«Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura».

questioni puramente tecniche. È ovvio che sembra incredibile dover parlare nel 2016 del reato di tortura per porre un divieto alla stessa. Dovremmo essere in una civiltà talmente avanzata che di tortura non se ne dovrebbe nemmeno parlare.

in un delitto di tipo naturale come la tortura. Le persone erano sottoposte a un insieme di sofferenze psichiche con totale annientamento della dignità della persona.

o una persona, come è successo, che piglia a martellate i passanti. Poi ci sono le situazioni in cui i cittadini, per difendersi, chiamano la polizia e i carabinieri che accorrono per difenderli.

Il problema è che quando in questo provvedimento parliamo di tortura confondiamo i piani. Che il povero Regeni sia stato torturato è chiarissimo

in tutti questi casi l'accusa era di atteggiamenti colposi!" Nel caso Uva sono stati assolti tutti: per tre volte il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione

aveva il viso gonfio e segni evidenti negli occhi, ma dal punto di vista fisico stava benissimo. Si muoveva e il fatto delle vertebre rotte assolutamente non sussisteva.

il povero Aldrovandi, in una situazione tale che gli avrebbe procurato l'infarto. Guardate che è esattamente la stessa identica cosa che è accaduta davanti a Palazzo Chigi, quando è stato colpito un carabiniere, da parte di un tale Preiti e i colleghi carabinieri invece di sparare all'aggressore gli sono saltati addosso e lo hanno buttato per terra. Andate a vedere tutte le foto con il carabiniere a cavalcioni dell'aggressore, che gli mette le mano dietro la schiena e le manette.

dovrebbero essere accusati di tortura. Credo che non ci sia mafioso o membro della 'ndrangheta che venga arrestato e interrogato in maniera ruvida, che non dirà immediatamente che è stato torturato,

la tortura? Su quale strada ci stiamo incamminando rispetto a chi deve intervenire per tutelare l'incolumità di tutti? Attenzione, mentre l'aggressore certamente commette un reato e mette in pericolo la vita dei cittadini, il carabiniere o il poliziotto devono intervenire, mettendo così a rischio la propria vita per difendere quella degli altri.

pregiudizialmente si accusano i poliziotti. L'avvocato Anselmo aggiunge - andate a leggere le interviste - che lui le cause non le vince in tribunale ma sui *media,* perché riesce a creare una pressione talmente grande sui *media* che comunque poliziotti e carabinieri, anche se non hanno fatto niente, stanno tre o quattro anni sotto processo. Si rovinano le loro vite, le loro famiglie vengono minacciate, le foto vengono messe sui *media*. Quando, poi, vengono assolti non serve a nulla, perché la professoressa Di Cesare, anche davanti ad una assoluzione passata in giudicato, dice che questi sono colpevoli di tortura.

modo teniamo aperte talune fattispecie nel nostro Paese. Io ho fatto il carabiniere di leva, ma non tutti hanno fatto il carabiniere di leva; hanno una storia diversa alle spalle rispetto alla concezione che hanno dei carabinieri e dei poliziotti. Certo, quando si dice che c'è una cultura di violenza nei carabinieri o nella polizia, e quindi pregiudizialmente si suppone che, quando questi intervengono, lo fanno esercitando questo tipo di violenza, benissimo, anzi malissimo: se lo fanno - e se viene provato - devono essere giudicati con la massima severità. Ma attenzione, pensiamo a quando un carabiniere o un poliziotto - cito ancora il caso davanti a Palazzo Chigi - interviene per bloccare una persona, specialmente se alterata. Basti pensare al caso Magherini: quante telefonate sono arrivate da cittadini perché quello aveva buttato una donna fuori da un taxi e aveva aggredito un'altra persona dentro: era nel classico delirio da cocaina. Fermare una persona così non è facile perché in questi casi quella mena, si ribella. Se succede qualcosa, se succede un imprevisto, cosa fa il poliziotto o il carabiniere? Sa già da prima che se interviene a bloccare una persona così rischia l'ergastolo? Non solo rischia la vita, ma rischia comunque di andare sotto processo? Sapete che persino nel caso Aldrovandi la Corte dei conti ha quasi annullato la sanzione rispetto a quei poliziotti dicendo che alla fine sono intervenuti come il regolamento imponeva loro di fare per bloccare una persona che resisteva all'arresto. Se tenendolo per terra in quella posizione, con le manette dietro la schiena, c'è stato un caso accidentale, non discuto. La sentenza c'è: omicidio colposo per negligenza, imperizia; lo hanno tenuto nella posizione sbagliata. Ma è forse tortura, come tutti vanno dicendo? Il problema è che l'Italia è uno strano Paese perché prima di fare una norma bisognerebbe mettersi d'accordo sulle finalità della stessa. Questo provvedimento serve se un caso Regeni succede in Italia, sia il canaro, sia un privato, quel tale che aveva preso prigioniero uno che lo prendeva in giro, e per una settimana a Roma lo ha torturato in tutte le maniere possibili e poi lo ha ucciso: certo che è giusto

Ma qui facciamo un'operazione pubblico-mediatica in cui indichiamo come tortura un certo tipo di comportamento. Volete che non ci sia preoccupazione nei poliziotti, nei carabinieri, nei capi della Polizia e dei Carabinieri che sono venuti in Commissione a spiegare

E, se questo avviene nel momento in cui i poliziotti intervengono, questi che fanno? Vanno all'ergastolo, perché sono colpevoli di essere intervenuti nel momento in cui è successo questo fatto, che sarebbe successo anche e comunque senza il loro intervento? per precisare meglio quello che vogliamo fare e lo facciamo alla luce di quello che insistentemente ogni giorno i *media*, e non solo i *media*, riportano. Se non fosse stato il «Corriere della sera», che è il maggiore giornale italiano, a dare cinque giorni fa fa un grande spazio a questo professore, indicando questi quattro casi di tortura, tutti colposi, che dovrebbero essere puniti come tali, noi non avremmo questa preoccupazione. Purtroppo l'aspettativa è quella e pertanto i nostri emendamenti sono volti a precisare ulteriormente le finalità di questo provvedimento.

Ma bisogna partire da un dato di fatto: nonostante la ratifica di numerose convenzioni internazionali, l'Italia ha finora disatteso l'obbligo di incriminare la tortura di tortura è considerato nel diritto internazionale una norma di diritto cogente, cioè inderogabile anche in situazioni d'emergenza, così come previsto dalla Convenzione siglata nel 1984 e recepita dall'Italia quattro anni dopo. Non solo, gli Stati devono anche esercitare una sistematica sorveglianza su regolamenti, istruzioni, metodi e pratiche di interrogatorio, nonché sulle disposizioni relative a custodia e trattamento di persone sottoposte in qualsiasi modo a limitazioni della propria libertà. dopo la ratifica della Convenzione contro la tortura, l'Italia non ha sentito la necessità di introdurre un reato *ad hoc*, perché si riteneva che nel nostro codice fossero già previste delle fattispecie idonee a punire tutti gli atti indicati nell'articolo 1, anche quelli commessi da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. Il nostro Governo sostenne tale posizione nei *report* inviati al Comitato contro la tortura nel 1990, nel 1994 e nel 1998. Solo nel *report* del 2002 le autorità italiane riconobbero espressamente la necessità di modificare le previsioni del codice penale. Il provvedimento, che dovrebbe recepire anche l'invito della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, è diventato ancora più urgente dopo la condanna ricevuta dall'Italia in merito alle torture commesse dalla polizia nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001. L'assenza di una fattispecie che permette di punire in modo proporzionato condotte particolarmente efferate poste in essere dalle Forze dell'ordine è stata infatti motivo di censura sia a livello internazionale, sia da parte dei giudici chiamati a decidere su quella vicenda, i quali hanno rilevato che le condotte inumane e degradanti accertate in giudizio avrebbero potuto indubbiamente essere ricomprese nella nozione di tortura prevista dalla Convenzione, denunciando così l'inadeguatezza delle fattispecie incriminatrici per cui gli imputati erano chiamati a rispondere. La *ratio* sottesa all'introduzione del reato di tortura può essere ricondotta a due ordini di considerazioni: da un lato, le informazioni estorte mediante tortura non possono essere ritenute attendibili per venire assunte come prova in un procedimento penale; dall'altro lato, la sanzione di inutilizzabilità dovrebbe rimuovere gli incentivi per l'utilizzo della tortura, contribuendo così a prevenirla. Ma è da marzo 2013 che è in atto un rimpallo sul testo tra i due rami del Parlamento. Al centro della questione c'è soprattutto la preoccupazione, sottolineata dai vertici di Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, che non si vada a configurare un reato contro le Forze dell'ordine. Dopo un primo testo approvato al Senato, poi ampiamente corretto dalla Camera, da quasi un anno il provvedimento è finito nel limbo, dopo il mandato al relatore conferito dalla Commissione giustizia Ora siamo tornati, con qualche correzione, al testo originario uscito dal Senato. Si contestualizza ciò che fa scattare la pena; viene introdotta l'espressione «reiterate violenze», l'agire «con crudeltà» e il «verificabile trauma psichico». Sul punto relativo alle Forze dell'ordine, torna la dicitura originale del Senato. Nel testo della Camera era invece specificato: «Se i fatti (...) sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni». Il testo che torna oggi nell'Aula del Senato prevede invece: «Se i fatti (...) sono commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni la pena è della reclusione da cinque a dodici anni». In poche parole, diminuiscono le sanzioni, e il reato, che rimane comune e non proprio di pubblico ufficiale, come è invece prescritto dalla Convenzione di New York, diventa ancora più generico. Affinché venga considerata tortura, per esempio, la violenza e la minaccia devono essere reiterate. Spariscono anche, tra le finalità elencate per definire meglio la fattispecie, quelle discriminatorie etniche, religiose o sessuali; così come sparisce la locuzione «per vincere una resistenza», accogliendo un rilievo mosso dal prefetto Pansa, secondo il quale per il testo della Camera poteva essere considerato un torturatore anche chi «causa una sofferenza acuta» (quindi anche con una singola manganellata), con il dolo specifico di «vincere una resistenza». Ma siccome il codice penale, all'articolo 53, stabilisce all'opposto che è compito del poliziotto «vincere una resistenza», si sarebbero profilati conflitti di giurisprudenza. I vertici delle Forze dell'ordine hanno in particolare messo l'accento sul rischio che con questa legge non si possa più garantire l'ordine pubblico, perché ogni tafferuglio potrebbe essere seguito da un diluvio di denunce alla magistratura. Si confrontano insomma due esigenze: la tutela dell'ordine pubblico e il rispetto dei diritti umani. E in questo senso è stato disperante ascoltare un procuratore generale della nostra Repubblica dire che Stefano Cucchi è stato vittima di tortura, come Giulio Regeni, quando era nelle mani dello Stato italiano. conclusione ritengo che difendere i diritti umani e rendere operative le Convenzioni internazionali contro la tortura non sia un atto contro qualcuno, ma un atto a garanzia di tutti, e che se anche questa legislatura si concludesse con un nulla di fatto sarebbe un fallimento che la politica non si può permettere. Signor Presidente, colleghe e colleghi, non vi nascondo il compiacimento personale nel potere intervenire quest'oggi sul provvedimento in esame. La proposta di legge, al di là dei giudizi dettagliati sul contenuto e dei singoli convincimenti, ha il merito di introdurre nel nostro ordinamento, nel codice penale, il reato di tortura. L'assenza nel nostro ordinamento di questo reato ha dell'incredibile, essendo l'Italia la Patria di Cesare Beccaria e di Pietro Verri, che oltre duecento anni fa avevano già trattato e stigmatizzato la pratica della tortura. Per la verità, la proposta di legge è stata contraddistinta da un *iter* legislativo molto difficile, a volte incoerente, ed i colleghi che mi hanno preceduto l'hanno già Eppure, su un tema così importante mi sarei aspettato una convergenza di posizioni che guardassero di più alla portata sociale e internazionale delle future disposizioni che a quella, molto più miope, della politica nazionale. Infatti, l'ordinamento italiano non prevede fattispecie in merito al delitto di tortura, nonostante la Costituzione, all'articolo 13, comma quarto, stabilisca che è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Resta il fatto che sia trascorso molto tempo da quando l'Italia, nel 1988, ha ratificato la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottata nel 1984 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 39/461. Non meno importanti, poi, sono i numerosi trattati e accordi internazionali che sanciscono che nessuno possa essere sottoposto a tortura, soprattutto se tra questi vi è la più volte citata Convenzione del 1984, che è quella che definisce, in maniera specifica, il reato in oggetto. Orbene, colleghi, concorderete con me che sia giunto il momento storico di dotare il nostro ordinamento di una figura di reato apposita, in maniera univoca e chiara, non solo perché è emerso dal dibattito pubblico quanto sia ormai necessario, ma soprattutto colmare un *vulnus* normativo non più accettabile. Lo dimostrano anche i recenti episodi di cronaca nei quali quei comportamenti criminosi sarebbero stati puniti in maniera più efficace e più puntuale qualora il nostro ordinamento fosse stato dotato di questo tipo di reato. Affermo e sottolineo quanto detto, perché noi non siamo solamente dei legislatori ma anche dei cittadini, che credono nella giustizia e - ancor di più - credono nella tutela dei diritti umani, in tutte le sue forme, soprattutto quelle più garantiste. Non occorre essere certo esperti giuristi o particolari promotori della dignità umana per attestare che, in materia, il nostro ordinamento è contraddistinto da un *deficit* di tutela. Basta leggere qualche pagina degli atti giudiziari su quanto accaduto tra il 19 e il 21 luglio 2001 a Genova in occasione del G8, oppure sui casi di Cucchi e Aldrovandi. Si tratta di vicende oscure che lasciano trapelare quel senso di inadeguatezza e incompletezza del nostro sistema penale nel reagire a violazioni sulla dignità di essere umano, nella sua integrità e perfino sulla vita. Come accennavo prima, l'*iter* legislativo è stato molto disordinato, e non posso non manifestare il mio disappunto sulla pretestuosa volontà da parte della Camera di stravolgere un provvedimento approvato all'unanimità in prima lettura al Senato, con nessuno voto contrario e tre soli astenuti.

cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, cura o assistenza. Ritengo si possa soprassedere sul ribadire quanto gravi debbano essere le minacce e quanto debbano essere reiterate le violenze. Forse è quel punto d'incontro tra varie posizioni che ci aiuterà ad andare avanti. L'articolo 613-*bis*, poi, contempla l'aggravante se l'autore del reato è un pubblico ufficiale, con una reclusione da cinque a dodici anni. Infine (aggiungerei finalmente),

delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura. Questo articolo rappresenta - a mio modesto parere - una tutela *a priori* per eventuali azioni coercitive avute con tortura al fine di ottenere dichiarazioni. Mi preme, tuttavia, sottolineare che il testo della Convenzione definisce la tortura come un comportamento che richiede il coinvolgimento di un pubblico ufficiale (o di chi esercita una pubblica funzione), chiarendo al contempo che eventuali definizioni più ampie non pregiudicano l'oggetto della norma. Tale è stata la soluzione accolta dal Parlamento, così giungendo ad un compromesso ragionevole tra posizioni altrimenti difficilmente conciliabili tra di loro, che avrebbero di fatto impedito l'introduzione di questa fattispecie di reato nel nostro ordinamento. Sinceramente, avrei personalmente preferito un recepimento quasi letterale del testo della Convenzione. Ad ogni modo, come anticipato precedentemente, ritengo importante si stia finalmente colmando una gravissima lacuna normativa e civile. Ciò detto, colleghi, vorrei però sottolineare una mia personale opinione ovvero che le disposizioni che stiamo introducendo nel nostro ordinamento penale non sono e non devono essere utilizzate in in modo strumentale per colpire le nostre Forze dell'ordine, che compiono il proprio dovere a difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini, operando molte volte nel rischio personale, nel pieno rispetto della legge e delle garanzie costituzionali dei cittadini. Quello che dobbiamo tenere ben presente è l'obiettivo della Convenzione di New York contro la tortura che era, ed è, prevalentemente diretto a quei Paesi che sono retti da regimi anti-democratici e che, per tale motivi, praticano largamente sui propri cittadini maltrattamenti fisici e di tortura. Detto questo, è evidente che le norme presenti nel nostro ordinamento, contro comportamenti assimilabili a pratiche di tortura, possono essere rafforzate ed è in questa logica che va valutato il voto che daremo a questo provvedimento. Concludendo, signor Presidente, introdurre il reato di tortura nel nostro codice penale significa non solo colmare una lacuna normativa particolarmente grave, ma significa smetterla di fare finta che il nostro Paese non abbia avuto episodi in tale senso. Qui stiamo trattando una questione che ha un enorme rilievo, soprattutto internazionale e deve essere affrontato e discusso come un passo avanti nella civiltà del popolo italiano. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo bene che ci sono le convenzioni e gli accordi internazionali, che sono stati più volte richiamati e che devono portare l'Italia ad adempiere a queste intese. Tuttavia, l'*iter*, anche complesso, di questa legge dimostra che le affermazioni che in molti passaggi, sia qui al Senato ma poi, successivamente, anche alla Camera, gli esponenti di Forza Italia hanno svolto hanno un loro fondamento. In molti casi, anche di fronte a fatti di cronaca che hanno causato sconcerto e a interrogativi in un senso e nell'altro, avendo assistito a processi mediatici, ad assoluzioni nelle aule di giustizia e a vicende che ovviamente hanno colpito tutti - l'epilogo tragico di vite è sempre una tragedia - non c'è dubbio che nell'animo di molti questa legge è stata più volte letta come un atto di diffidenza, e non vorrei dire di ostilità - ma potrei anche dire di ostilità - nei confronti delle forze di polizia. L'uso legittimo della forza è un tema delicato, sia nell'ambito dei trattati che delle intese dell'ONU. Si attua una norma costituzionale. L'Italia ripudia la guerra, ma ovviamente, se le organizzazioni internazionali - ed è successo nel corso della storia, anche recente hanno deciso di contrastare dittature, invasioni e decimazioni di popoli, ha partecipato a iniziative di siffatto tipo, dove si ritiene che ci sia un uso legittimo della forza, anche quella militare più estrema. E così nel campo dell'ordine e della sicurezza pubblica sono chiamate a operare le forze di polizia, talvolta anche le Forze armate, che vengono utilizzate pacificamente, spesso per presidiare

Diciamo che poi non accade nulla, perché - per fortuna - la deterrenza esercitata dalla presenza e dal controllo del territorio fa sì che quei soldati che vediamo, anche uscendo qui dal Senato, all'angolo di San Luigi dei Francesi o a piazza Cavour, davanti al Palazzo di giustizia, poi non usino legittimamente la forza, perché nessuno li costringe a questo, ma sono lì perché, in teoria, ciò potrebbe accadere. E, quindi, sia le forze di polizia che le Forze armate hanno questo diritto. È ovvio che la tortura, di cui si parla, non è consentita a nessuno e nemmeno l'uso legittimo della forza ammette le vessazioni e le prepotenze. Dopo di che c'è un'area grigia

ai danni di persone in stato di fermo o di detenzione, che quindi sono affidate all'autorità pubblica, che può trattenerle in attesa dell'accertamento di responsabilità. Se poi c'è una condanna, le può trattenere a maggiore ragione per l'espiazione della condanna, ma quella persona già viene trattenuta e non può essere sottoposta a una vessazione, meno che mai a una violenza. Per questo già numerose norme consentono nel nostro ordinamento d'impedire l'arbitrio i reati - ne posso fare un elenco sommario - di percosse, lesioni, violenza privata, minacce, ingiurie, sequestro di persona o arresto illegale, con tutte le sanzioni previste per l'indebita limitazione della libertà personale, l'abuso di autorità nei confronti di arrestati o detenuti, perquisizioni o ispezioni personali arbitrarie. Insomma, il nostro codice presenta una gamma di norme e sanzioni che impedisce, appunto, l'arbitrio. Ciò è tanto vero che le vicende evocate, compresa quella di Genova, hanno visto, in assenza di questo reato, processi, condanne estromissioni - poi il tempo ci dirà se giuste o sbagliate - anche di altissimi dirigenti delle nostre forze di polizia. Quindi, non è che in assenza di questa norma c'è il libero arbitrio, ci sono la violenza di Stato e la tortura. Se diciamo questo, facciamo un grave errore.

Il nostro Gruppo interverrà e ci sono ancora emendamenti che abbiamo presentato. Richiamo una particolare attenzione ai temi della sicurezza e delle forze di polizia e conservo un fondo di perplessità maggiore di altri, perché diffido delle intenzioni di alcuni. il combinato disposto della norma sulla tortura e quella che non è stata fatta sui numeri di identificazione delle forze di polizia non vorrei che portasse a una paralisi delle azioni di ordine pubblico, perché poi nell'azione di ordine pubblico l'Italia negli ultimi mesi non ha vissuto momenti allarmanti, ma potrebbero esserci. È infatti anche tutti i temi del degrado della vita nelle città, spesso connessi al dilagare dell'immigrazione clandestina o della criminalità comune, in alcuni quartieri si collegano anche all'ordine pubblico. Spesso si tenta di impedire l'arresto di esponenti della criminalità organizzata in alcune parti d'Italia, e non solo in quelle in cui mafia, camorra e 'ndrangheta sono più forti; è successo anche a Roma.

Non so se si usino più la fascia tricolore e lo squillo di tromba, ma, colleghi, attenzione a non favorire in maniera esagerata le denunce arbitrarie.

che vengono dalla Commissione giustizia sono spesso oggetto di lunga discussione in quest'Assemblea e spesso sono anche motivo di un'inevitabile discussione, per via dell'imprecisione di alcune decisioni, che abbiamo visto, anche recentemente,

per introdurre quella ragionevolezza sulla differenza tra gli abusi, che non devono essere effettivamente commessi, e l'uso legittimo della forza a tutela della legalità, dell'ordine pubblico, dell'esecuzione di un ordine di arresto nei confronti della camorra. I limiti sono molto labili.

anche nella scorsa legislatura, quando ero Capogruppo, abbiamo rafforzato ulteriormente il 41*-bis* perché la magistratura di sorveglianza e l'ordinamento giudiziario avevano chiesto una maggiore e più precisa definizione delle norme, per evitare il collegamento dall'interno all'esterno. A volte anche quello che può sembrare vessatorio (il vetro

la loro catena di comando. Ma, nell'ambito delle norme che ho già citato, ritengo questa norma - con buona pace dei trattati internazionali - ultronea. Può servire a combattere la tortura in quei Paesi assolutisti, nelle dittature, dove peraltro se ne fregano delle convenzioni internazionali, le calpestano e fanno di tutto e di più, e questo non è accettabile.

venga la pausa di riflessione che è durata molto a lungo, per evitare una paralisi dell'azione di sicurezza e di contrasto anche per quanto riguarda le espulsioni e quant'altro, visto che il testo è stato in parte modificato. Qualcuno dice che non si può fare l'espulsione, a parte che il Governo si occupa più dell'ingresso e del trasporto dei clandestini.

quarta. Evidentemente l'adempimento dei trattati internazionali non è scevro dalla saggezza del legislatore. Tutti siamo contro le torture e le violenze, ma è bene avere a mente l'uso legittimo della forza, la possibilità di mantenere l'ordine pubblico, il non scoraggiare il personale delle forze di polizia che già è scontento per i contratti, per il riordino delle carriere,

alla riflessione cui il Senato ha contribuito, sta contribuendo e contribuirà, perché il testo arrivato dalla Commissione avrà ulteriori modifiche. Io ho presentato emendamenti che mi auguro vengano approvati. Il relatore ha dato un contributo e mi auguro che ciò possa indurre anche la Camera e tutto il Parlamento a una riflessione. La tortura va combattuta. La forza della legalità non va paralizzata.

coerentemente con quanto contenuto nei trattati internazionali ai quali abbiamo aderito e cui facciamo riferimento.

Cosa non ci convince? L'ha detto prima benissimo il senatore Manconi. Non ci convince l'idea che sta alla base del testo che è stato così fortemente ridimensionato introducendo formule come «reiterate violenze» e «minacce gravi», cambiando la natura del reato di fatto un concetto di crudeltà che a noi pare assolutamente privo di senso in ragione del reato e del delitto che si intende punire. La tortura di per sé prevede la crudeltà. Non c'è bisogno di una specificazione.

e, soprattutto, a un certo tipo di Stati. Non a caso in questo Senato, pochi giorni fa, si è svolta una grande discussione su un emendamento che tutti abbiamo definito emendamento Regeni. Uno Stato autoritario, colpevole di un'azione nei confronti di un cittadino italiano, innocente sotto ogni profilo, ha utilizzato la tortura nell'idea di estorcere informazioni con la violenza. Cosa c'è di più crudele della consapevolezza di utilizzare uno strumento di violenza verso una persona per estorcere informazioni o per imporre comportamenti? Ogni specificazione è particolarmente incomprensibile perché sembra difensiva. È una sorta di *excusatio* *non* *petita*. Siccome penso che si possa verificare nell'ambito dei comportamenti dello Stato, anche del nostro Stato,

vogliamo difendere le migliori condizioni di vita che abbiamo conquistato. Noi tutti riteniamo che le libertà personali siano qualcosa di sacro che non possiamo in modo assoluto mettere in pericolo. Noi tutti sappiamo

del porto di Buenos Aires, andato in Argentina con la famiglia per lavorare, che si è fatto strada nella sua attività,

buttato vivo da un aereo, così come si usava fare nei confronti degli oppositori di quel regime fascista.

ambiguo, nascosto e vigliacco. Il reato di tortura va introdotto come riconoscimento doveroso e come come atto di condanna nei confronti di queste modalità di agire degli Stati. i nostri operatori: anzi, sono convinto del contrario. Quando dico che non c'è bisogno di giustificarsi, dico che siamo convinti che i nostri operatori, gli operatori delle Forze dell'ordine e della giustizia, hanno in sé così maturato lo spirito democratico e il rispetto dei diritti dell'uomo che non sono interessati, se non in una deviazione episodica

vorrei iniziare con una citazione. Nel 1972 Carlo Alberto Dalla Chiesa disse: «L'Italia può sopravvivere alla perdita di Aldo Moro all'introduzione della tortura». In queste semplici parole c'è l'enunciazione assoluta e condivisibilissima dell'incompatibilità tra tortura e democrazia. Il reato di tortura, insomma, è la più grave forma di degenerazione di un'autorità in violenza, di un potere in arbitrio. L'introduzione di questo reato è attesa persino da troppi anni nel nostro ordinamento, ed è tanto più necessario e urgente farlo adesso, ora, alla vigilia del *referendum* sulle riforme costituzionali più dannoso della storia della Repubblica. un motivo in più, insomma, per fare presto; un motivo che si aggiunge alla necessità di assolvere agli obblighi cui il nostro Paese è notoriamente inadempiente da oltre trent'anni. Nel merito delle modifiche intervenute in Commissione giustizia al Senato, rilevo che sono state in buona parte da noi condivise. Il testo pervenuto dalla Camera andava necessariamente cambiato. Noi alla Camera ci eravamo astenuti su quel testo, nonostante fossimo e siamo tuttora tra i più convinti assertori della necessità di introdurre questo reato nel nostro ordinamento. Ci eravamo astenuti perché quel testo introduceva limiti probatori molto difficili per l'accertamento del reato, con la prevedibile conseguenza che sarebbe stato, appunto, difficoltoso, se non addirittura impossibile, in sede processuale, pervenire all'accertamento del reato di tortura. Mi riferisco nel dettaglio alla necessità di dimostrare l'intenzionalità delle condotte. Nel caso, per esempio, di Federico Aldrovandi, non c'è dubbio alcuno che vi sia stata tortura, essendo stato vittima di ben 54 ripetuti atti di violenza. Ma ben difficilmente si potrebbe dimostrare l'intenzionalità nell'infliggere tortura.

È di tutta evidenza che non potrebbe essere che così, ma tale prova addizionale renderebbe più complesso l'accertamento del fatto da parte del magistrato. Ancora, si sarebbe dovuto accertare se la persona torturata fosse stata affidata al suo torturatore, ovvero sottoposta alla sua autorità, vigilanza e custodia: elementi difficilmente dimostrabili, anche in un caso conclamato come quello dei ben noti fatti accaduti alla Diaz. A queste criticità - segnalate dal Movimento 5 Stelle alla Camera - la Commissione giustizia del Senato ha opportunamente risposto modificando il testo modificando il testo in maniera sostanziale. Rimangono, tuttavia, anche altre criticità, a cui si potrebbe agevolmente porre rimedio semplicemente recuperando i nostri emendamenti. Non convince - ad esempio - il termine «reiterate» riferito alle violenze e alle minacce gravi. È notorio, infatti, che l'articolo 1 della Convenzione ONU sulla tortura riferisce al singolo atto di violenza. modo, non convince il termine «verificabile» riferito al trauma psichico, per cui al danno per le vittime di violenza seguirà l'umiliazione di una visita con lo psichiatra. Chiediamo inoltre che anche i trattamenti inumani o degradanti la dignità umana debbano essere inseriti nel novero dei comportamenti suscettibili di rappresentare reato di tortura. Ricordo che questa previsione era stata peraltro già oggetto di approvazione da parte della Commissione giustizia del Senato e anche dall'Assemblea del Senato nella precedente lettura. Infine, se non vogliamo che vadano ad aggiungersi anche i procedimenti per tortura al novero degli oltre 1,5 milioni di processi prescritti dall'entrata in vigore dall'ex Cirielli, dev'essere opportunamente considerato il raddoppio dei termini di prescrizione. In conclusione, dobbiamo fare una legge giusta, necessaria e urgente, ma dobbiamo anche fare una legge che sia efficace. Per questo motivo, invito tutti, Governo, Assemblea, relatori, a guardare con particolare attenzione alle criticità evidenziate. Peraltro - come ho già detto - sarebbero facilmente superabili con l'accoglimento degli emendamenti presentati dal nostro Gruppo, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame non può più permettersi ulteriori correttivi e, quindi, ulteriore *navette* tra Camera e Senato. Di tempo ne è già passato fin troppo. Adesso è arrivato il momento, al contrario, di accelerare e lo dobbiamo fare per Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, Aldo Bianzino,

Senatore Giovanardi, per cortesia, ciascuno, se non eccede, può dire quello che vuole. Il giudizio spetta poi a coloro che ascoltano, sia all'interno di quest'Aula

MPL))*. Gentile Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione sulla scomparsa di Sisinio Zito, che per ben cinque legislature ha animato i lavori di quest'Assemblea, rappresentando magistralmente la Calabria. Il senatore Zito, originario della bellissima Roccella Jonica, nel corso della sua lunga carriera politica è stato più volte Sottosegretario, nonché Presidente della Commissione sanità del Senato Politico scafato e calabrese orgoglioso, non ha mai lesinato giudizi e consigli, sempre saggi e puntuali. Indimenticabile il suo impegno come sindaco di Roccella Jonica, città che ha valorizzato con iniziative dall'altissimo valore culturale e sociale, rendendola una vera e propria perla della costa reggina e di tutto il Mediterraneo. Il suo impegno come politico e amministratore deve essere di esempio per tutti coloro i quali intendono fare del proprio territorio l'unica ragione della loro attività politica. A tutta la famiglia di Sisinio Zito esprimo il mio affetto e la mia sincera vicinanza e lo faccio in quest'Aula dove, per molto tempo, il senatore Zito ha fatto sentire la sua voce, contribuendo ad animare i lavori parlamentari.

Grazie,

che, nelle prossime settimane, potranno ricevere una lettera di licenziamento. Non dobbiamo arrivare a questo, lavorando tutti insieme per trovare una soluzione, così come avvenuto in altre Province italiane. Penso alla Sicilia, alla Calabria

Signor Presidente, poco fa al Senato della Repubblica, a pochi metri da quest'Aula, nella sala Koch, si è tenuto il XVII evento annuale della multinazionale Ericsson. Il titolo scelto per l'iniziativa è: «Giovani, innovazione, crescita», titolo nobile e incoraggiante. Peccato che in Italia la Ericsson, in questi giorni, stia facendo tutto il contrario. Con che coraggio si può parlare di giovani, innovazione e crescita, quando il 13 giugno scorso, negli stabilimenti Ericsson, è stata aperta una procedura di mobilità per 302 lavoratori e 30 dirigenti? E questo per il 2016, più altri 53 entro i primi sei mesi del 2017. Complimenti per il concetto di sviluppo! Da diversi anni Da diversi anni Ericsson non ha un piano industriale neppure a medio termine per l'Italia. Ericsson ha aperto ben 13 procedure di mobilità dal 2007 ad oggi e continua a disinvestire in ricerca e sviluppo nel nostro Paese. L'azienda sta mettendo in ginocchio moltissimi lavoratori qualificati e preparati. E noi mettiamo loro i tappeti rossi? Caso emblematico è il centro di ricerche di Pisa, nella mia Toscana, dove gli obiettivi strategici sono proprio quelli di sviluppare nuovi concetti di sistema, testare nuove tecnologie, nonché sviluppare prototipi di sistemi avanzati. Là la mattanza, signor Presidente, è già iniziata. Per affrontare la crisi aziendale apertasi in Ericsson, è stato proposto un Il Vice Ministro dello sviluppo economico, la signora Teresa Bellanova, con sicurezza scriveva su Twitter: «Il tavolo sulla crisi di Ericsson è convocato al MISE per mercoledì 22 giugno». Un'azienda seria si sarebbe resa ovviamente disponibile. Tuttavia, i vertici dell'azienda hanno stracciato l'impegno, hanno pensato bene di snobbare i lavoratori e le istituzioni italiane, facendoci sentire una loro colonia. È un caso molto grave, uno smacco alle istituzioni nazionali e regionali coinvolte e soprattutto un grave affronto ai lavoratori, che da anni, con il loro lavoro, contribuiscono al successo di

e l'accesso ai fondi europei (quello sì, lo sanno fare bene). Dopo aver investito nel nostro Paese, Ericsson sta gradualmente, ma inesorabilmente ridimensionando la propria presenza in Italia. In questa situazione, signor Presidente, che trovo molto grave mi dissocio da chi pensa di poter utilizzare le istituzioni come una passerella o come *location* per i propri eventi. Palazzo Madama è innanzitutto la casa dei cittadini italiani. Presidente, non siamo ancora una colonia delle potenze economiche mondiali. Per cortesia, lo riferisca al signor Renzi e al senatore Napolitano. *(Applausi dal Gruppo che ha disertato la riunione del MISE, è un fatto molto grave. Ma ancora più grave è il comportamento di chi, come vice presidente del Senato Gasparri e il ministro Poletti, hanno aperto le porte di Palazzo Madama ai vertici Ericsson senza valutarne le conseguenze. La prossima volta vadano davanti agli stabilimenti, con di fronte i lavoratori in mobilità, e annuncino, come pochi minuti fa ha dichiarato la ministra Giannini, che è in previsione di inglobare, nel prossimo futuro, il 5 per cento di tirocinanti, probabilmente usa e getta. Vedremo poi se i lavoratori saranno contenti di essere licenziati per dar posto e acquisire nuova forza lavoro al minor prezzo e a minori tutele. Licenziano 385 persone persone con contratti dignitosi, per riprenderne 200 usa e getta. Signor Presidente, come sempre questo Governo si dimostra per quello è: debole con i forti e forte con i deboli. Renzi, stai sereno. *(Applausi